Colleghi, visto che non ci sono proprio le folle, questa mattina, cerchiamo almeno di ascoltarci, così si dà la conferma ad un vecchio proverbio, se non altro.

*relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 996, molto simile al n. 747 (di cui difatti si propone l'assorbimento nel primo), si prefigge l'obiettivo di sancire l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, una istituzione culturale o da altri soggetti stranieri, durante la loro temporanea permanenza in Italia, perché siano esposti al pubblico nel corso di eventi Durante l'esame in 7a Commissione, a questo disegno di legge, composto da un solo articolo, è stato presentato e approvato un articolato emendamento, che contribuisce a meglio definirne il testo. Le grandi, prestigiose mostre sono occasioni uniche, spesso indimenticabili, storiche, non solo per gli studiosi, ma anche per il vasto pubblico di visitatori, italiani e stranieri, per approfondire la conoscenza dell'arte, che si tratti di un singolo artista, ovvero di grandi e complessi movimenti artistici. Il Trecento, Giotto e le influenze bizantine, il Rinascimento, Caravaggio e i caravaggisti, Bernini e il barocco, Canova e il neoclassico, l'impressionismo, il futurismo, l'astrattismo, il surrealismo e, poi, l'arte antica greca e romana, le grandi stagioni artistiche orientali, con i tesori dell'arte cinese e indiana, la ricostruzione di importantissime collezioni, come la Giustiniani che, qualche anno fa, fu esposta proprio a Palazzo Giustiniani, o quella Farnese, ora in mostra all'Ambasciata di Francia. Certo, non tutti i capolavori italiani sono rimasti nel nostro Paese: molti sono disseminati nei musei e nelle collezioni pubbliche e private, così come le opere degli artisti stranieri che, in occasione di mostre prestigiose, devono essere reperite nel mondo intero. Le mostre costituiscono importanti operazioni culturali, scientifiche, divulgative e sono motivo di attrazione per centinaia di migliaia di visitatori e turisti. Queste iniziative sono state fino ad oggi ostacolate dalla indisponibilità di alcuni prestatori stranieri ad inviare opere in Italia, perché non vi era la certezza della restituzione, a causa di potenziali provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Vorrei sottolineare, quanto alla compatibilità compatibilità delle disposizioni del disegno di legge, che esse non si applicano ai beni che costituiscono corpo del reato, qualora il reato sia stato commesso in Italia. Inoltre iniziative legislative analoghe sono state già adottate in altri Paesi europei, come Francia e Germania, oltre che negli Stati Uniti. Assume in merito un valore emblematico il caso delle opere d'arte presenti a Taiwan nel museo di Taipei, testimonianze eccezionali dell'antica civiltà cinese che le autorità taiwanesi raramente, e solo con espresse garanzie di restituzione, hanno prestato a Paesi esteri, in quanto il Governo taiwanese teme che la Repubblica popolare cinese, reclamante la proprietà delle opere, possa chiederne il sequestro quando esse sono presenti nel territorio di altri Stati. Questo è anche il caso di opere italiane all'estero. Un esempio per tutti: la celebre biga etrusca di Monteleone di Spoleto, unica al mondo, esposta al Metropolitan Museum of Art di New York, non è mai stata prestata e non è mai tornata nel nostro Paese. Al fine di superare il rischio-sequestro, che limita concretamente la circolazione delle opere d'arte nel mondo, la presente proposta è volta a garantirne e assicurarne la restituzione alle istituzioni che le hanno messe a nostra disposizione, indipendentemente dalla natura e dallo stato di eventuali controversie sul diritto di proprietà. Inoltre viene attribuito al Ministero degli affari esteri e al Ministero per i beni e le attività culturali un ruolo preminente, riconoscendo loro il potere di predisporre, con apposito decreto, in occasione di ogni esposizione, la lista delle opere d'arte ottenute in prestito, che sono insequestrabili, la durata del prestito e i responsabili delle esposizioni che si assumono l'impegno alla restituzione del materiale ricevuto.

mentre quello oggi in discussione ha ottenuto il parere favorevole del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, come ha riferito il sottosegretario Giro durante l'esame in sede referente. Raccomando perciò vivamente all'Aula l'approvazione del provvedimento, che in 7ª Commissione ha registrato il consenso unanime di tutte le forze politiche.

della relatrice, senatrice De Feo, che ringrazio. Questo disegno di legge rappresenta un contributo alla diffusione della cultura, alla circolazione ed alla conoscenza delle opere d'arte nel nostro Paese. Come la relatrice ha sottolineato, spesso si crea un blocco alla completezza di una mostra per paura del sequestro di opere d'arte che sono oggetto di contenzioso tra Stati o istituzioni. Si tratta non di rado di veri propri capolavori che vengono preclusi alla circolazione, che non vengono prestati al nostro Paese per non correre il rischio, appunto, del sequestro. Come ha sottolineato la senatrice De Feo, altri Paesi, come la Francia e la Germania, ma anche gli Stati Uniti, si sono già dotati di una legislazione sulla certezza della restituzione di opere d'arte contese e prestate per mostre temporanee. Questo disegno di legge garantisce la certezza della restituzione a quelle istituzioni che le hanno messe a disposizione degli organizzatori delle varie mostre. Ciò peraltro - questo va sottolineato - senza compromettere eventuali indagini sul diritto di proprietà. Viene inoltre previsto - e questo ci convince molto - un ruolo di garanzia del Ministero, che viene ad avere un duplice ruolo. Innanzitutto, si prevede che il Ministero possa predisporre la lista delle opere d'arte date in prestito e dichiarate insequestrabili, almeno nel periodo di durata dell'evento. In secondo luogo, il testo iniziale del disegno di legge è stato ulteriormente migliorato grazie a un emendamento del Gruppo del Partito Democratico presentato in Commissione, a prima firma del senatore Marcucci, che prevede, proprio a maggiore garanzia dei prestatori di opere d'arte, che il Ministero dia l'autorizzazione all'organizzazione dell'evento, sulla base di una domanda dei soggetti che intendono organizzarlo. Quindi, vi è una piena condivisione del Gruppo del Partito Democratico su un disegno di legge i cui contenuti sono all'attenzione del Parlamento da più legislature. Ci auguriamo vivamente che almeno in questo

Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la relatrice, senatrice De Feo, che con impegno è riuscita a portare avanti questi due disegni di legge, uno a prima firma del senatore

che firmatario del disegno di legge nella legislatura precedente è stato il senatore Gustavo Selva, certamente persona di grande rilievo e di grande spessore culturale, che si era fortemente impegnato nell'approvazione della legge stessa. Quindi, sono lieta che oggi si possa giungere ad una conclusione positiva, perché il fatto che l'intera 7a Commissione abbia inteso votare i testi concordati indica un atteggiamento comune nei riguardi di un disegno di legge che, in fin dei conti, rappresenta la necessità, da parte dell'Italia, di colmare un vuoto normativo. Che si tratti un vuoto normativo è da rilevare rispetto a quanto già ricordato, cioè alle norme che già esistono, ormai da diverso tempo, da decenni, in alcuni Paesi, come

che ha una legge che risale al 1998. Già questi Paesi si erano posti il problema della insequestrabilità delle opere d'arte, e non è un fatto secondario, perché le opere d'arte appartengono al patrimonio culturale dell'umanità, non a questo o a quel Paese. Starei per dire, senza retorica, ma con preciso convincimento, che la conoscenza delle opere d'arte contribuisce molto a creare dei rapporti, che partono dall'ambito culturale e tra le diverse espressioni sociali dei diversi Paesi del mondo e contribuiscono anche a creare un'atmosfera di pace, di serenità e di rispetto della dignità delle culture degli altri.

di carattere culturale. Questa è un'iniziativa che può sembrare quasi secondaria, ma che secondaria certamente non è, perché contribuisce a rendere comune il patrimonio culturale dell'umanità. Noi siamo lieti che, anche da parte del Governo, ci sia stata una espressione di volontà positiva nei riguardi di questo testo concordato, così come emendato, come ricordava anche la collega Franco, dal Gruppo del Partito Democratico, e quindi con una condivisione comune. È importante sottolineare anche il ruolo che il Ministero per i beni e le attività culturali assume nell'ambito di questo testo, proprio con l'iniziativa di determinare una lista di beni, che rappresenta un dato oggettivo di riferimento nel momento in cui si deve poi applicare la norma stessa. Mi sia consentito, al termine di questo breve intervento, oltre a ringraziare ancora una volta

nella città di Castellaneta in Puglia. Grazie all'intervento immediato del sottosegretario Villari si è creato un tavolo di concertazione che, a proposito di cultura della pace,

se il Sottosegretario o il Ministro vorranno venire direttamente sul luogo per constatare l'importanza della scoperta e per assicurare l'intervento del Ministero, affinché pubblico e privato possano lavorare insieme al recupero di una zona archeologica di particolare pregio. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, il disegno di legge in titolo si propone di superare i limiti alla circolazione dei beni nel mondo, assicurando l'insequestrabilità delle opere prestate all'Italia e la loro restituzione, indipendentemente dalla natura e dallo stato di eventuali controversie sul diritto di proprietà. Il disposto relativo all'insequestrabilità dei beni si applica solo nei casi in cui non siano applicabili convenzioni, accordi internazionali o norme comunitarie. In questo modo viene garantito che l'attuazione delle disposizioni in oggetto non risulti in contrasto con gli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia. Inoltre, tale disegno di legge non importa una deroga a principi sostanziali e procedurali del diritto penale, in quanto essi non si applicano ai beni che costituiscano corpo di reato, qualora il reato sia commesso in Italia. Si specifica, inoltre, che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie e, in particolare, in caso di sentenza definitiva, resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca. Si sottolinea che l'Italia ha sempre contrastato illeciti in materia di importazioni, esportazioni e trasferimento di proprietà dei beni culturali ed ha conseguentemente sottoscritto e ratificato accordi internazionali che permettono non solo di agire per la restituzione di opere d'arte illegittimamente uscite dal territorio italiano, ma anche di assicurare il ritorno in altri Stati di beni culturali rubati o illecitamente esportati. Le conquiste e i progressi compiuti nel nostro Paese in difesa del patrimonio artistico si ravvisano nel primo provvedimento organico di tutela: n. 364 del 20 giugno 1909. Uno dei punti fondamentali della legge del 1909 è il riconoscimento del prevalente interesse pubblico delle opere d'arte e d'antichità, enucleando i principi dell'inalienabilità per le cose appartenenti allo Stato e agli enti pubblici insieme al divieto di esportazione, qualora questa costituisca un danno per la storia e l'arte della nazione, principi poi ribaditi dalla Costituzione. Infatti, nel 1948 l'importanza della tutela, insieme alla promozione e alla conoscenza del paesaggio e del patrimonio storico artistico, fu dettata dall'articolo 9 della Costituzione repubblicana. A livello europeo, invece, una serie di convenzioni internazionali suggerivano norme per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Ai regolamenti si affiancò, nel secondo Novecento, una significativa presa di coscienza da parte della collettività, scaturita sull'onda emozionale della ricostruzione, dei restauri e dei recuperi dei beni trafugati durante la guerra. In seguito, episodi come la straordinaria impresa degli «angeli del fango», accorsi da tutto il mondo per salvare i tesori di Firenze, inondata dall'alluvione del 1966, hanno contribuito a scrivere importanti pagine della storia della tutela. Tornando all'attualità, si ricorda la Convenzione dell'UNIDROIT, ratificata in Italia con la legge 7 giugno 1999, n. 213, finalizzata ad ottenere la restituzione di beni culturali rubati e di quelli illecitamente esportati, nonché il decreto legislativo n. 42 del 2004, che recepisce la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, la quale legittima i vari Stati membri dell'Unione europea all'azione di restituzione, al fine di recuperare i beni illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro e presumibilmente presenti nel territorio italiano. Emblematico è il caso delle opere artistiche conservate presso il Museo nazionale di Taipei, che rappresentano capolavori purtroppo raramente esposti all'estero. Soltanto in quattro occasioni quei capolavori sono stati esibiti in Europa (a Parigi, a Berlino, a Bonn e a Vienna) per non sottometterli al rischio che Pechino ne chieda il sequestro. Si tratta di una quantità di eccezionali testimonianze dell'antica civiltà cinese che solo chi si reca a Taiwan può ammirare. Questa è la ragione per la quale, in Italia, non è stato finora possibile organizzare una mostra nonostante la disponibilità offerta dalle competenti autorità taiwanesi.

non solo nello specifico caso di Taiwan. Sulla base di tali disposizioni sono stati realizzati, nei citati Paesi, grandi eventi espositivi, che hanno avuto un'ampia risonanza anche internazionale, e che non è possibile replicare nel nostro Paese in mancanza della disciplina che si prefigge di introdurre il Il provvedimento sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e l'impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa, anche giudiziaria, promossa da chiunque: Paese estero o istituzioni pubbliche e private. A tal fine, il disegno di legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e al Ministro per i beni e le attività culturali un ruolo preminente, riconoscendo loro il potere di predisporre, in occasione di ogni esposizione, con apposito decreto, la lista delle opere d'arte prestate ed insequestrabili, oltre la durata del prestito e l'indicazione dei responsabili delle esposizioni. esposizioni. Concludo affermando che si tratta di un'iniziativa legislativa lodevole. Lo scambio culturale di opere d'arte unisce popolazioni di tutto il mondo per mezzo dell'instaurazione di un dialogo continuativo tramite l'arte, elemento essenziale della nostra società, che adempie al suo ruolo, oltre che estetico, psichico, pulsionale, di valore essenziale nell'identità dell'uomo. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, che ha visto in Commissione la condivisione *bipartisan* di maggioranza e opposizione, ha lo scopo di favorire lo scambio di opere d'arte tra i musei di tutto il mondo senza il pericolo del possibile sequestro delle stesse, l'esemplificazione - il caso del Museo nazionale di Taipei - e, soprattutto, l'offerta ad un più vasto pubblico della possibilità di ammirare questi capolavori.

di esporre in Italia quei capolavori italiani oggi disseminati in tutto il mondo in collezioni pubbliche, e soprattutto - ne possiamo capire le difficoltà ancora più evidenti - in collezioni private.

Signor Presidente, saluto con viva soddisfazione l'arrivo in Aula del disegno di legge del collega Malan, di cui sono cofirmatario, relativo alle disposizioni in materia di non sequestrabilità di opere d'arte prestate al nostro Paese - da uno Stato, da un museo o da un ente culturale straniero - in temporanea esportazione per essere esposte in Italia, nel corso di eventi di interesse culturale ed artistico. presente disegno di legge - che era già stato proposto nella XIV e XV legislatura, da numerosissimi colleghi senatori e deputati di ogni schieramento parlamentare, e che era stato già approvato nel 2006 dalla Commissione cultura della Camera, non riuscendo a terminare l'*iter* legislativo in Aula - viene a colmare un evidente vuoto normativo che ha finora impedito al nostro Paese di ospitare mostre di capolavori d'arte provenienti da Stati, musei o enti stranieri non disponibili a prestarli, in assenza di una certezza giuridica che ne garantisse la restituzione al soggetto prestatore. Il testo normativo che ci accingiamo a votare è pienamente integrato e complementare con tutte le normative vigenti - nazionali ed europee - relative alla tutela dei beni culturali e con le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia per il contrasto e la repressione dei traffici illeciti in questo campo; esso, inoltre, ha ottenuto il parere favorevole del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Abbiamo proposto questo provvedimento (che è stato oggetto dell'intelligente lavoro dei colleghi della 7a Commissione e della relatrice, senatrice De Feo, che ringrazio) ispirandoci alle analoghe leggi già da molti anni in vigore in Paesi quali l'Austria, la Francia, la Germania e gli Stati Uniti, al fine di garantire e assicurare la restituzione delle opere d'arte alle istituzioni che le hanno messe a nostra disposizione, indipendentemente dalla natura e dallo stato di eventuali controversie sul diritto di proprietà e attribuendo al Ministero degli affari esteri e al Ministero per i beni e le attività culturali un ruolo preminente nella gestione del prestito e nella restituzione delle stesse opere. Il provvedimento consentirà, finalmente, di organizzare anche nel nostro Paese - come è già avvenuto, con grande successo, nelle Nazioni testé citate - importanti mostre di meravigliose opere d'arte di plurimillenaria antichità, come quelle esposte nel Museo nazionale di Taipei, a Taiwan: avori, bronzi, coralli, giade, pitture e porcellane che attirano ogni anno milioni di visitatori. Penso anche all'opportunità che avremo, allo stesso modo, di ammirare splendidi capolavori russi e di altri Paesi che l'Italia non ha mai potuto ospitare *pro-tempore* proprio per il vuoto legislativo che oggi, con questo provvedimento necessario, andiamo definitivamente a colmare.

abbiano problemi di rivendicazioni. Il senatore Zanetta l'ha già ricordato: Taipei, per quanto riguarda la Cina popolare, ma anche le nuove Repubbliche nate dalla disgregazione dell'impero russo. In ogni caso, si tratta di Paesi di nuova costituzione dove il patrimonio non ha ancora una certezza, e pertanto le nuove amministrazioni hanno la tendenza ad evitare

per meglio definire e approfondire i limiti e le applicazioni della normativa, che tratta una questione molto delicata. Voglio anche ricordare come nelle due precedenti legislature, prima alla Camera e poi al Senato, questo provvedimento

Voglio altresì sottolineare, ed è utile portare di ciò a conoscenza l'Assemblea, come la normativa in questione garantisca in pieno l'applicabilità delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e come il Ministero si sia premurato di acquisire il parere del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in ordine a un eventuale impatto negativo sulle funzioni di tutela, che è stato assolutamente scongiurato. per la delicatezza della materia, ringrazio ancora la relatrice e la Commissione, che in maniera unitaria ha svolto un lavoro egregio. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo».

per l'importante lavoro svolto. È importante ricordare che il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare e anche quello assorbito erano tra i lavori della nostra Commissione già dal 2009 e, nonostante numerose calendarizzazioni garantite dal collega Possa, presidente, sono occorsi ben due anni per l'approvazione di un testo sul quale, peraltro, si è ottenuto il consenso unanime dei Gruppi. È evidente che quando c'è la volontà di raggiungere un risultato, questo lo si ottiene, ed è altrettanto evidente che forse avremmo potuto raggiungerlo prima. Ricordo, inoltre, che siamo ancora all'approvazione di un solo ramo del Parlamento e speriamo che possa seguire rapidamente anche quella dell'altra Camera. Il disegno di legge in questione, come abbiamo avuto modo di apprendere durante i lavori, detta disposizioni certe sui modi con i quali le opere d'arte, di proprietà di altri Paesi o enti, debbano circolare nel nostro Paese. In altre parole, questo disegno di legge sancisce la certezza che le opere prestate al nostro Paese non siano oggetto di esercizio di ulteriori diritti, quali il sequestro conservativo da esplicarsi sulle opere stesse. il disegno di legge restringe la limitazione alla insequestrabilità solo alle opere sulle quali sia in corso un contenzioso sulla proprietà. Sappiamo tutti come le grandi esposizioni artistiche, frutto dello scambio delle opere d'arte tra i musei dei vari Paesi del mondo, costituiscano uno dei più importanti mezzi di promozione e diffusione della cultura e rappresentino per il pubblico un'occasione unica ed irripetibile per ammirare, apprezzare e conoscere opere di altissimo valore artistico, storico e culturale. Avere dunque la possibilità di ricevere opere d'inestimabile valore al fine di poterle esporre al pubblico nel corso di eventi d'interesse culturale e artistico, incrementandone la circolazione, è un traguardo al quale il nostro Paese, dato il valore delle opere d'arte detenute, sarebbe dovuto arrivare già da qualche tempo. Lo scambio delle opere d'arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è certamente uno dei mezzi fondamentali per promuovere la diffusione della cultura, un modo per garantire la conoscenza al pubblico, un modo per riuscire a mettere insieme in una sola mostra i tanti capolavori sparsi per il mondo. Il principio che si vuole affermare è che i cittadini devono poter usufruire del diritto di ammirare capolavori che rappresentano un patrimonio dell'umanità. Questo provvedimento sancisce perfettamente l'insequestrabilità dei beni prestati e contestualmente l'impegno alla loro restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa giudiziaria promossa da Paesi esteri

preminente all'interno della procedura prevista per il rilascio della lista delle opere d'arte ottenute in prestito, che sono insequestrabili, riportando anche la durata del prestito e i responsabili delle esposizioni che si assumono l'impegno alla restituzione del materiale ricevuto. Per questi motivi, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori

Il disegno di legge in esame - che ha l'obiettivo di stabilire l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un'istituzione culturale o da altri soggetti stranieri, durante la loro temporanea permanenza in Italia per essere esposte al pubblico nel corso di eventi d'interesse culturale e artistico - è estremamente importante e arriva ben dopo quello che hanno fatto anche altri Stati europei. Le grandi e importanti mostre espositive che avvengono nel nostro Paese da sempre sono una grande attrattiva per milioni di visitatori sia stranieri che italiani. non tutti i capolavori italiani sono rimasti nel nostro Paese, com'è già stato evidenziato dalla relatrice: molti sono disseminati nei musei e nelle collezioni - pubbliche, ma anche private - di tutto il mondo. Uno per tutti è la nostra Gioconda di Leonardo da Vinci, che troneggia nel famosissimo Museo del Louvre di Parigi, ugualmente sparse in tutto il pianeta sono le opere di artisti stranieri che in occasione di mostre prestigiose fatichiamo spesso a reperire. Un dato inconfutabile è che le mostre e le esposizioni in genere sono a tutti gli effetti una una straordinaria occasione di richiamo sia di turisti sia di visitatori, che esse garantiscono al nostro Paese notevoli entrate di carattere economico e che rappresentano momenti di grande arricchimento culturale, perché consentono uno scambio, un dialogo tra i popoli, grazie a linguaggio universale che è quello dell'arte. Lo scambio di opere d'arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi più importanti ed efficienti per la diffusione della cultura, al quale, soprattutto negli ultimi tempi, si ricorre con frequenza sempre maggiore. Ciò ci consente di organizzare mostre di grande interesse, non solo per gli studiosi, ma anche per un vasto Riunire in una sola rassegna capolavori sparsi in diverse parti del mondo può diventare un'occasione irripetibile per consentire anche a grandi masse la fruizione di opere d'arte meravigliose, che hanno la valenza di edificarci culturalmente e spiritualmente e soprattutto hanno una grande valenza educativa e pedagogica: anche chi non è in grado di viaggiare, infatti, può così essere messo in condizione di partecipare a questi momenti eccezionali per allargare anche i confini delle proprie conoscenze. È evidente, quindi, la notevole valenza delle disposizioni recate nel presente disegno di legge, che si pone nella giusta direzione di assicurare la diffusione della cultura, dando al grande pubblico la possibilità di ammirare opere d'arte di altissimo pregio, di grande valore storico e artistico, sovente sottratte invece alla circolazione internazionale proprio a causa della paura che alcuni Paesi ed istituzioni hanno del pericolo di non vedersele restituire, una volta che le hanno cedute soltanto temporaneamente. infatti di trovarsi di fronte a fortissime difficoltà nel reperire questo materiale artistico da altri Paesi, in quanto da parte loro si teme proprio per la loro restituzione.

Il presente disegno di legge è volto a garantire ed assicurare la restituzione delle opere alle istituzioni che le hanno messe a nostra disposizione, indipendentemente dalla natura e dallo stato di eventuali controversie sul diritto di proprietà, perché spesso questo è uno dei punti dirimenti. Con esso, viene inoltre attribuito al Ministero degli affari esteri e al Ministero per i beni e le attività culturali un ruolo preminente, riconoscendo loro il potere di predisporre, con un apposito decreto, in occasione di ogni esposizione, la lista delle opere d'arte che sono state ottenute in prestito, che diventano così insequestrabili, la durata del prestito e i responsabili delle esposizioni, che si assumono l'impegno alla restituzione del materiale ricevuto. In virtù di quanto sopra detto non posso che esprimere il convinto voto favorevole del mio Gruppo.

il disegno di legge in titolo contribuisce a incrementare la collaborazione tra istituti museali e culturali internazionali, ai fini dell'accrescimento della qualità dello scambio e dell'offerta culturale nel suo complesso. Le mostre internazionali costituiscono un importante strumento di valorizzazione del nostro patrimonio. A seguito dell'azione prodotta dal «Gruppo Bizot», composto dai direttori dei grandi musei d'arte europei e nordamericani, scaturito nella pubblicazione dei «Principi generali per la gestione dei prestiti e lo scambio di opere d'arte tra istituzioni culturali», il tema della mobilità delle collezioni d'arte è stato affrontato in modo sistematico a livello europeo. Il primo risultato è stato il documento «*Lending to Europe*» (2005), un insieme di linee guida che intendevano orientare l'azione di musei, Stati membri e istituzioni europee verso l'individuazione dei modi e degli strumenti atti a facilitare per il futuro il prestito di collezioni museali su scala europea. Si sono successivamente costituiti gruppi di lavoro incaricati di mettere a punto soluzioni operative per i seguenti temi: amministrazione dei prestiti e standard di prestito; sistemi di garanzia statale; valutazione, autoassicurazione, rinuncia all'assicurazione; compensi per il prestito e prestiti a lungo termine; costruzione dei rapporti di fiducia e lavoro in rete; e infine il principio, oggetto del disegno di legge in discussione, la garanzia di non sequestrabilità. Emblematico è il caso delle opere artistiche conservate presso il Museo nazionale di Taipei, che rappresentano capolavori purtroppo raramente esposti all'estero (soltanto in quattro occasioni quei capolavori sono stati esibiti in Europa: a Parigi, a Berlino, a Bonn e a Vienna) per non sottometterli al rischio che Pechino ne chieda il sequestro. Questa è la ragione per la quale da noi non è stato finora possibile organizzare una mostra, nonostante la disponibilità offerta dalle competenti autorità taiwanesi. Come sottolineato dal relatore, per superare tale ostacolo e favorire al contempo la tutela delle opere a rischio di sequestrabilità, gli Stati Uniti d'America con legge n. 898-259 del 1965, la Francia con legge n. 94-679 del 1994, la Germania con legge del 1998 e l'Austria con legge sullo sviluppo economico e sulla competitività del 2003, hanno garantito la restituzione delle opere d'arte prestate da istituzioni museali e culturali, senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle controversie sul diritto di proprietà. La presente proposta colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del moltiplicarsi, specie dopo i rivolgimenti dell'ultimo decennio, di situazioni come quella di Taiwan. Essa sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e l'impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque: Paese estero o istituzioni pubbliche e private. Ovviamente è stato introdotto un limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai principi di diritto penale, specificando che esse non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso nel nostro Paese. Si specifica, inoltre, che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili, proseguono secondo le procedure ordinarie e, in particolare, in caso di sentenza definitiva resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca. Dichiaro dunque il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

le grandi esposizioni culturali sono ormai un volano fondamentale del nostro turismo. In una stagione come la nostra, attraversata da una domanda crescente di *short break*, le mostre d'arte sono un fattore determinante della mobilità turistica. È un settore sempre più emergente che si contraddistingue per l'elevato grado di internazionalità, per il medio-alto potere d'acquisto dei fruitori e per il basso peso della stagionalità. Tre requisiti fondamentali per un Paese come il nostro che può vantare un numero davvero imponente di città d'arte e di itinerari culturali. In tale contesto, la competitività tra le città europee viene giocata anche e soprattutto sulla capacità di organizzare grandi mostre e grandi eventi culturali. Ecco perché è determinante affrontare e risolvere la questione della circolazione delle opere d'arte e la pratica dei prestiti museali. la ringrazio - nel presentare il disegno di legge, sull'Italia pesava l'indisponibilità di alcuni importanti prestatori stranieri ad inviare opere nel nostro Paese, a causa dell'incertezza della restituzione per eventuali provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Con questo provvedimento in titolo vogliamo garantire le istituzioni internazionali che mettono a nostra disposizione le opere d'arte per mostre temporanee, svincolando totalmente tale procedura dallo stato di potenziali controversie sul diritto di proprietà. In modo particolare, voglio sottolineare la centralità del Ministero dei beni e le attività culturali, così come avevamo espressamente richiesto anche attraverso un emendamento presentato dal Gruppo del Partito Democratico in 7a Commissione, poi sottoscritto anche dal Gruppo dell'Italia dei Valori; dovrà predisporre per ogni mostra la lista delle opere ottenute in prestito, la durata del prestito e l'impegno alla restituzione nei modi e nei tempi concordati con le istituzioni proprietarie dei beni. È quindi con soddisfazione che il Gruppo del Partito Democratico esprime un voto favorevole su tale disegno di legge che contribuisce al rafforzamento dell'offerta culturale italiana, assicurando al mercato dell'arte internazionale un provvedimento che stabilisce la certezza dei prestatori stranieri sulla restituzione delle opere d'arte concesse. D'altra parte così è stato fatto negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e in Austria. La cultura e la sua diffusione sono e rimarranno priorità del Partito Democratico.

abbiamo il tempo sufficiente per realizzare finalmente un desiderio di tutta la cittadinanza italiana - il Parlamento è l'espressione di tutta la cittadinanza - e spero quindi che ciò avvenga.

voglio sottolineare l'importanza di questo provvedimento, ringraziare per l'ottimo lavoro svolto la relatrice e tutti i senatori e le senatrici della 7a Commissione,

e migliorare la collaborazione sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione dell'atto mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e avrà un'azione stabilizzatrice di una particolare area, di valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale. L'Accordo è composto da 17 articoli. Per l'articolo 1, le Parti agiranno in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per sviluppare la cooperazione, basandosi sul principio della reciprocità, e potranno stipulare eventuali accordi tecnici. L'articolo 2 individua i campi e le forme di cooperazione.

La ringrazio, signor Presidente. L'articolo 4 stabilisce che venga costituita una commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione. L'articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attività militari. L'articolo 6 riguarda il rilascio dei visti richiesti dal personale militare. L'articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell'espletamento delle sue funzioni. L'articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospitante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera. L'articolo 9 prevede che, in caso di infrazioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verrà escluso dagli *stage* e dai corsi di addestramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. dispone che il personale interessato si conformerà alle direttive delle autorità militari dell'ente ospitante. L'articolo 11 stabilisce che, in caso di assenza illegale di un membro del Paese inviante sul territorio dello Stato ricevente, le autorità di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle autorità del Paese di origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo. L'articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati. L'articolo 16 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali. L'articolo 17 regola l'entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e le modalità di recesso. Quanto al disegno di legge, esso reca l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la copertura finanziaria pari a circa 10.000 euro l'armo, ad anni alterni, in relazione allo svolgimento in Marocco delle riunioni della commissione mista. Ricordo peraltro come, nel corso della presente legislatura, il Parlamento abbia già approvato due autorizzazioni alla ratifica di Accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, in particolare in materia di sistema globale di navigazione satellitare e di trasporto aereo. Richiamo nuovamente il buon andamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati, le quali hanno costituito un importante fattore di stabilizzazione e dialogo tra l'Europa e il mondo arabo. Ricordo peraltro come l'Accordo in esame, al di là del contenuto proprio e del fatto che fu sottoscritto nel 2006 in un contesto geopolitico del tutto diverso da quello odierno, giunga oggi all'esame dell'Aula nel momento in cui il Mar Mediterraneo è al centro dell'attenzione per le vicende tunisine, egiziane e oggi libiche. Nel contesto attuale la vicenda del Marocco si sta mantenendo su caratteri peculiari, poiché vi sono state manifestazioni nei confronti del Re e del Governo, ma finora la situazione (anche per il profilo riformista e moderno del monarca Mohammed VI) risulta sostanzialmente tranquilla. Sarebbe ascrivibile al nuovo corso riformatore anche la decisione del Re, del 14 aprile 2011, di concedere la grazia a 190 detenuti per reati politici. Fra di essi, in particolare, vi è anche un attivista saharawi, che è stato liberato, e un connazionale, Abdelkrim Britel, condannato per associazione eversiva. Decisiva è stata anche l'azione di mediazione posta in essere dal neocostituito Consiglio nazionale dei diritti dell'uomo e dal suo segretario generale, Mohamed Sebbar. Non dobbiamo inoltre dimenticare che il 28 aprile scorso un brutto attentato ha colpito la città di Marrakech, provocando decine di vittime (e quindi anche in questo caso noi esprimiamo piena solidarietà al Marocco e alla città di Marrakech). Incerto risulta essere il movente di tale attentato, anche se pare sia ascrivibile a posizioni integraliste che vogliono forse rallentare il processo di modernizzazione e il nuovo corso avviato in Marocco. Per il Marocco, così come per gli altri Stati dell'area, al di là dei Governi in carica, è essenziale il dialogo con l'Europa. Ed è interesse primario dell'Italia e degli altri Stati membri dell'Unione europea favorire tale processo. In tal senso, ogni Accordo stipulato con Paesi sinceramente impegnati nella costruzione di relazioni euro-mediterranee sempre migliori, finisce con l'avere senz'altro un'utilità di carattere politico che travalica il loro stretto contenuto. In conclusione, per tutte queste motivazioni, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

sponda Sud del Mediterraneo, che in questo momento sono attraversati da forti tensioni e turbolenze che promettono un'evoluzione democratica, ma che naturalmente comportano in questa fase delle problematiche non di poco conto sul terreno del rapporto tra società civile e regimi politici quanto alla capacità dei regimi politici stessi di favorire un'evoluzione democratica dei loro Paesi, che invece spesso vediamo essere spinti sulla linea assolutamente sbagliata e inaccettabile di una reazione forte, in alcuni casi brutale, contro le loro popolazioni e in aperta e a volte gravissima violazione dei diritti umani. È il caso della Libia, che sappiamo essere ancora attraversata da un conflitto nel quale anche il nostro Paese è coinvolto, e poi, andando verso Est, è il caso molto grave dello Yemen, della Siria. Insomma siamo in un contesto di grande delicatezza. Il Marocco ha scelto una strada positiva, una strada di dialogo per le riforme e quindi di una transizione morbida verso la democrazia. ci auguriamo, e faremo di tutto - credo - come Paese perché questa strada venga portata avanti con determinazione, con decisione e con equilibrio. Il Marocco ha anche un'antica questione aperta e irrisolta, ossia quella che riguarda lo statuto, il futuro del Sahara occidentale, che sappiamo essere conteso, con un forte movimento indipendentista, che è stato sempre sostenuto anche dalle risoluzioni delle Nazioni Unite; vi è un contenzioso aperto, perché in questo momento c'è un'occupazione da parte del Marocco del Sahara occidentale. È in corso un negoziato molto delicato che è avviato su una strada positiva, che noi incoraggiamo, che credo che il Paese, l'Italia, il Governo italiano stia incoraggiando e debba incoraggiare. Tuttavia, è una ferita aperta, è un problema aperto nel Marocco. con un Paese che sta evolvendo in modo positivo, che è nel pieno di una transizione democratica positiva e di un processo di negoziato di pacificazione con il popolo saharawi, ma appunto, data la delicatezza di questi temi, credo sia opportuno e necessario, da parte del nostro Paese, avere un'attenzione e anche un elemento di cautela. È per questa ragione che abbiamo presentato l'ordine del giorno

per il Sahara occidentale, «sia nei contatti bilaterali che in sede europea o in ambito ONU, affinché la questione del Sahara occidentale sia affrontata e risolta con il dialogo politico e il negoziato diplomatico, nel rigoroso rispetto dei diritti umani e dei diritti dei popoli». si impegna il Governo «a invitare le autorità marocchine a mantenere e rafforzare la scelta della via del dialogo per le riforme e del negoziato sotto egida ONU sulla questione del Sahara occidentale, anche come base per l'ulteriore sviluppo», che noi auspichiamo, naturalmente, «della collaborazione in ambito militare». Infine introduciamo una clausola: impegniamo il Governo «a ricorrere agli strumenti di natura diplomatica e giuridica, incluso l'avvio della procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo,» (quindi è una procedura prevista dall'Accordo)

di un Trattato internazionale. C'è un precedente importante che ha riguardato la ratifica di un Accordo di cooperazione con la Repubblica popolare cinese in campo culturale, in particolare cinematografico. Sappiamo che la Cina fa sistematico ricorso alla censura, e questo è un problema dal nostro punto di vista. Allora noi abbiamo pensato che fosse giusto accompagnare il sì alla ratifica di un Accordo - che comunque aiuta l'evoluzione nei rapporti positivi tra i popoli e quindi anche lo scambio culturale ed indirettamente l'apertura delle società con le quali entriamo

ci siano violazioni dei diritti umani, in questo caso del diritto umano fondamentale alla libertà di espressione. Ecco, noi abbiamo utilizzato questo precedente per applicarlo anche in questo Trattato, ovviamente su una fattispecie completamente diversa, cioè la cooperazione militare, che non può in nessun caso, qualora sfortunatamente

riserva di procedere alla denuncia di cui all'articolo 17, qualora la situazione dovesse prendere una strada negativa, oggi per la verità non prevedibile, oltre che non auspicabile. Concludo, dicendo che

abbiamo visto, nel caso totalmente diverso della Libia, cosa è derivato dal giusto e sacrosanto Accordo di amicizia italo-libica, che è un Accordo tra

il dialogo e il confronto tra i popoli; tuttavia, la mancanza di una clausola di denuncia ha reso delicata la posizione dell'Italia nei confronti della Libia. Allora io penso che questo elemento, la clausola di la clausola di denuncia, debba essere sempre presente nel trattati internazionali che l'Italia stipula, in generale e in modo particolare quando si tratta di Paesi che sono in una situazione di evoluzione, di transizione democratica e, come per tutte le transizioni, esposti

la grande attività, nel processo di amicizia e di cooperazione con il Regno del Marocco, svolta dalla nostra Associazione parlamentare, così come anche quella svolta pregevolmente su iniziativa di ISIAMED, l'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo, che grazie anche alla forte collaborazione e alla forte iniziativa dell'ambasciatore dell'ambasciatore del Marocco in Italia, Abo Ayoub, muove i primi passi e, congiuntamente all'associazione parlamentare, promuove tutte le iniziative utili a quel processo che il senatore Tonini ha prima di me illustrato.

altri importanti accordi bilaterali sono intercorsi tra il nostro Paese e il Marocco. Buon ultimo, l'ultimo accordo di cooperazione militare suggella un percorso già avviato sul piano culturale, sul piano della cooperazione istituzionale e sul piano economico, che è così importante. Lo sviluppo del Marocco è sotto gli occhi di tutti. Ricordo solo che oggi, in quel grande bacino del Mediterraneo, dove il dialogo e i ragionamenti tra una sponda e l'altra saranno capaci di determinare una nuova economia (che proprio nella culla del Mediterraneo affonda le sue radici), il porto di Tangeri è uno dei più importanti per la logistica internazionale e fa da specchio alle grandi iniziative della logistica italiana. italiana. Molte imprese italiane in Marocco trovano oggi le condizioni per poter sviluppare al meglio la loro iniziativa in cooperazione con le imprese e l'economia marocchina, e questo grazie al fatto che un processo di riforme, sia istituzionali che di altra natura, è stato avviato con coraggio dal Marocco, fin dai lontani anni '60. '60. Questo sovrano illuminato ha consentito al proprio popolo di percorrere la strada difficile della conquista della democrazia nei vari aspetti della vita economica e sociale. Un po' alla volta, si è compiuto questo piccolo e faticoso miracolo della condivisione e della libertà, della libertà, che il Marocco ha affrontato con tanto impegno. Noi non possiamo che valorizzare il più possibile questa esperienza, soprattutto nel momento in cui analizziamo il contesto che circonda il Marocco e l'esplosione avvenuta in questi ultimi mesi in quella parte del mondo così delicata e così strategica per gli equilibri del resto Vale dunque la pena di aggiungere alla ratifica di questo Accordo tutta la nostra adesione e tutto il nostro impegno convinto a favore del popolo marocchino, che insieme a quello italiano può giocare un ruolo importantissimo nella determinazione dei futuri equilibri di questo Mediterraneo, che deve poter continuare a crescere nel nome della democrazia, che non so se - come molti di noi sono convinti - sia un concetto esportabile. Certo, può essere una "malattia" contagiosa e può contagiare quindi quindi i Paesi confinanti con il Marocco, in un processo democratico lento ma che, inesorabilmente, dovrà avanzare. Lascio al senatore Adragna le conclusioni più significative di questa nostra collaborazione e della valorizzazione della ratifica di questo Accordo, come degli altri. alle riforme istituzionali importanti che hanno condotto il Marocco a conquistare grandi spazi nel sistema economico internazionale, ve ne è una che forse aiuterà più di tutte per il problema del Sahara occidentale e del del deserto, che prima il senatore Tonini citava. Aver concesso in questi anni, con un processo vero di *devolution* sostanziale sul modello catalano,

il processo autentico che il Governo marocchino e il Re del Marocco hanno compiuto in questi anni verso la democrazia sostanziale e formale.

Credo che con il voto di oggi l'Aula del Senato compia anche un significativo e forte gesto politico. Di fronte ai rivolgimenti che stanno avvenendo nella sponda Sud del Mediterraneo, noi, con questo che tocca la delicatissima materia della cooperazione militare, vogliamo con chiarezza manifestare una profonda e convinta fiducia verso un Paese amico. Il Marocco sta dimostrando, in effetti, seppur in coerenza con le sue tradizioni, di dare una risposta forte alle istanze che animano questa "primavera araba",

non è stata però di chiusura, di resistenza corporativa, ma di rilancio più profondo e complessivo del processo di revisione delle istituzioni marocchine. Dopo un fondamentale discorso del Sovrano alla Nazione, nel marzo scorso, si sta consolidando quel processo di riforma cui si faceva riferimento e che ha riguardato anche il diritto di famiglia e che ora sta riguardando i principi essenziali dell'assetto costituzionale, un processo che si dovrà concludere con un *referendum* popolare che proprio in questi giorni riguarderà un'organica Il primo pilastro di questa riforma è la costruzione di un vero sistema regionale, fondato su governi locali rappresentativi, dotati di una vera autonomia politica. In questa prospettiva, credo che, così come è negli auspici dell'ordine del giorno presentato da alcuni colleghi, si potrà trovare una soluzione soddisfacente alla storica questione del Sahara occidentale. Il secondo pilastro è quello del rafforzamento delle istituzioni rappresentative centrali nei confronti del potere monarchico. Guardate, a 150 anni dall'Unità del nostro Paese sembra di intravedere in Marocco un'evoluzione come quella che portò le istituzioni del Piemonte sabaudo a trasformarsi da una monarchia costituzionale in un vero e proprio sistema parlamentare. Queste riforme sono poi accompagnate da un rafforzamento dell'autonomia del potere giudiziario e, più in generale, del sistema della tutela dei diritti. nel leggere la complessa realtà degli eventi che si stanno svolgendo di fronte a noi nella sponda Sud del Mediterraneo dobbiamo essere capaci di apprezzare fino in fondo la risposta che viene dal Marocco, dal suo Governo e dalla sua classe politica, una risposta che, radicandosi nella storia di una monarchia più che centenaria, cerca di costruire una vera e radicale svolta democratica nella continuità istituzionale. Con questi sentimenti di fiducia verso un Paese amico e con la convinzione di dare oggi, anche con questo atto, un contributo concreto alla costruzione di un Mediterraneo più unito,

per i progressi significativi registrati sia nel settore sociale che nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A questo punto mi preme evidenziare, anche su sollecitazione degli intervenuti, in particolare del senatore Tonini, la delicatezza

nel valutare come estremamente importante per il nuovo equilibrio che si sta delineando in quella regione del mondo il ruolo che il Regno del Marocco può assolvere, è molto attento

questi accordi hanno una loro valenza e noi intendiamo affermare con certezza come la direzione di marcia debba essere parallela a quella del rispetto pieno dei diritti dell'uomo.

come segue: «a valutare l'opportunità di ricorrere agli strumenti di natura diplomatica e giuridica, incluso l'avvio della procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo, qualora vengano riscontrati, da parte delle competenti autorità marocchine, comportamenti che violino i diritti umani e le libertà fondamentali». PRESIDENTE. Chiedo

quelli già firmati con altri Stati in materia di cooperazione militare e anche di tutela e di autotutela. Tengo a sottolineare che è un momento delicato e, quindi, è significativa la ratifica che noi ci accingiamo ad

che non mi pare sia stata sottolineata abbastanza, della commissione mista per promuovere la cooperazione: si tratta di uno strumento che abbiamo sperimentato con successo in altri rapporti bilaterali e che - anche questa volta - credo e spero possa svolgere il ruolo che ha svolto in

C'è la Grecia che sta bruciando, per precise responsabilità di quella cricca finanziaria che governa i destini del mondo, coloro che fanno parte del Gruppo Bilderberg e anche coloro che si riuniscono in segreto per decidere dove mandare la speculazione. E allora, per fortuna domenica e lunedì anche i giovani italiani si sono cominciati a ribellare si sono raggiunti, dopo 16 anni, i *quorum*: 27 milioni di italiani hanno votato sui *referendum* contro la privatizzazione dell'acqua, contro l'energia nucleare e sul legittimo impedimento. mentre il Paese soffre, abbiamo un Governo e un Ministro dell'economia che vanno a braccetto con i banchieri. Cito, signor Presidente, un articolo di Nicola Borzi, che non è certo un bolscevico, ma scrive per «Il Sole 24 ORE». Cosa dice questo articolo? che il potere contrattuale dei banchieri in un'economia stagnante è predominante e si è talmente rafforzato, nei confronti delle istituzioni e della clientela, da vedere le banche protagoniste di importanti scelte di politica economica ed industriale. le intese con Governo e Confindustria. E a farne le spese chi sono? I consumatori, i risparmiatori, le famiglie, i clienti del credito al consumo.

vi furono il treno contro l'usura della Confesercenti e la Chiesa cattolica che si impegnò - e si aumentano i tassi di interesse sui mutui fino all'80 per cento. Capisco perché certe volte il Governo non risponde alle mie interrogazioni.

come Bisignani, che fa parte della cricca che arriva fin dentro i Palazzi del potere. Su Finmeccanica, sulla cricca di Bertolaso, e quant'altro, ho 30-40 interrogazioni parlamentari, senza ottenere alcuna risposta. Mi auguro che si cominci a rispondere, perché questo è un Paese dove c'è una generazione perduta che non ci perdonerà:

ma adesso c'è una generazione perduta. Noi facciamo da ammortizzatori sociali per i giovani, per una generazione di precari, ma un Governo che obbedisce alle richieste dei banchieri che futuro darà ai propri giovani?

ma il ministro Tremonti aveva detto che i banchieri o andavano in galera o venivano licenziati, e nessuno di loro è stato licenziato; è stato cacciato Profumo dai compagni di merende, però con 40 milioni di euro di buonuscita. Bisogna rispondere delle malefatte anche in Parlamento: è un dovere morale.